Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato oggi per le ore 13,30, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale». Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

al Documento di programmazione economico-finanziaria con cui si impegnava il Governo a procedere ad un ridimensionamento del numero dei Ministri e dei Sottosegretari in ragione del risparmio di spesa. Esso fu respinto in quella sede

la volontà di fare le cose, si fanno e basta, senza nascondersi dietro criteri di inammissibilità che servono solo a mascherare questo mastodontico Governo. Al momento, il riferimento alla decisione della 5a Commissione per me è scontato, obbligatorio e sono d'accordo con quanto ha fatto.

Signor Presidente, colleghi, vi è un quadro della finanza pubblica favorevole. E non capita spesso. Non sempre, infatti, siamo così fortunati da poter gestire un risultato positivo come quello dell'assestamento 2007, che oggi è sottoposto all'approvazione del Parlamento. Questo assestamento effettua la ricognizione della gestione, adeguando le dotazioni di carattere discrezionale in funzione dell'effettivo andamento della gestione amministrativa e delle relative esigenze. abbiamo a che fare con un assestamento nel quale il saldo, al netto delle regolazioni contabili e compreso l'impatto degli atti amministrativi, si colloca intorno ai 18,8 miliardi, rispetto alla previsione iniziale di 23 miliardi di euro. Un assestamento, quindi, nel quale si rileva un miglioramento del saldo netto di 4,2 miliardi di euro da finanziare in termini di competenza. Questo permette, pur nel rispetto del percorso di risanamento dei conti pubblici, di indirizzare risorse per l'adozione di un provvedimento volto, da un lato, al sostegno delle categorie sociali più deboli con l'adeguamento delle pensioni minime e, dall'altro, al finanziamento di interventi atti a favorire lo sviluppo. In questa situazione, anche grazie ad un più favorevole gettito tributario, per consentire alla pubblica amministrazione di poter perseguire i propri scopi più efficacemente nei settori cruciali della scuola, della sicurezza e nel contrasto all'evasione fiscale. Per tali motivi, noi del Gruppo Misto-Popolari-Udeur esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in oggetto.

richiamandomi alle motivazioni espresse in sede di discussione generale. Vorrei utilizzare il tempo a mia disposizione per affrontare due questioni che mi sembrano rilevanti e che già sono

parlamentari, non solo dell'opposizione, ed anche istituti accreditati ed economisti più o meno indipendenti si chiedono come mai l'Italia non abbia proceduto in questa direzione nell'anno 2007 e nelle previsioni dell'anno 2008.

credo che tale dato non possa essere contestato. Secondo l'impostazione più rigorista (se posso utilizzare questo termine), nonostante l'aggiustamento dell'1,3

il Governo abbia lavorato correttamente e nella direzione giusta, che rispettiamo ampiamente il Patto di stabilità interna

Governo. Queste maggiori entrate sono dovute non tanto alla politica antievasiva quanto agli anticipi di cassa, agli anticipi delle spese, all'IRPEF versato con le nuove assunzioni frutto della riforma Maroni.

colleghi, l'assestamento di bilancio di cui si discute contiene l'aggiornamento a metà esercizio degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto al 31 dicembre 2006. Con il decreto-legge n. 81, approvato nel luglio scorso, abbiamo già focalizzato molti aspetti critici sull'uso delle variazioni sul lato delle entrate derivanti dal maggiore gettito tributario. In quella sede ho anche evidenziato la discutibile procedura seguita: legiferare su una previsione di entrata non legittimata da una formale variazione di bilancio, così come si sta facendo, ma che doveva essere precedente al citato decreto-legge n. 81 e non successiva. Ciò detto, emerge comunque l'inadeguatezza dell'assestamento nella sua collocazione temporale rispetto ai valori corrispondenti agli andamenti di finanza pubblica. Si pensi, per esempio, al dato relativo all'autoliquidazione delle imposte sui redditi, che quest'anno è stato differito al 9 luglio - quindi, a dopo il 30 giugno, data di presentazione dell'assestamento che ha forte incidenza sulla quantificazione complessiva delle entrate. È di tutta evidenza come, anche sul lato della spesa, si abbiano conseguenti ripercussioni, oltre che contabili anche sociali e politiche, che l'assestamento non riesce a cogliere. Quindi registreremo, anche quest'anno, una successiva variazione di bilancio, stante la registrazione di un ulteriore extragettito. Speriamo che questa volta non ci sia un altro tesoretto da spartire, ma si migliorino i saldi di finanza pubblica, vera emergenza del Paese. In questo provvedimento, il saldo netto da finanziare migliora di oltre 4 miliardi, registrando sul fronte delle entrate un extragettito di 7 miliardi e 403 milioni, al netto dei 900 milioni dell'emendamento del Governo risalente al 26 settembre scorso, e con 5 miliardi derivanti da imposte dirette.

Nel 2007 è cresciuto il peso delle imposte dirette, quelle pagate dai cittadini contribuenti, rispetto al 2006 per colpa della finanziaria 2007 del Governo di centro-sinistra. Questo assestamento è la certificazione dell'aumento delle tasse degli italiani sui redditi. Ciò non ha niente a che fare, come ricordava qualche settimana fa il collega Baldassarri, con il maggiore gettito da recupero da evasione fiscale, e ciò per due motivi. *In primis*, le misure antielusione e antievasione di Visco non hanno finora potuto esplicare la loro efficacia. In secondo luogo, tali misure erano indirizzate soprattutto al lato della lotta all'elusione IVA e di altre imposte indirette rappresentanti appena 2 miliardi e 365 milioni della quota di extragettito complessiva, cioè meno di un terzo. Un altro dato preoccupante, rilevato sul lato della spesa, è l'aumento del costo degli interessi per il debito pubblico, aumentano per un miliardo e 365 milioni di euro in conto competenza. Indubbiamente, l'andamento del tasso di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea ma non è escluso che ci sia un aumento dell'indebitamento rispetto al tendenziale. L'aumento di 0,4 per cento a causa del tesoretto ha comportato una rivisitazione in aumento sia del debito pubblico che del disavanzo con conseguente ricaduta negativa sul costo degli interessi. Il debito pubblico, e i suoi costi, sono la tassa peggiore che passiamo alle future generazioni senza che questo Governo faccia niente. Dal lato della spesa pubblica, inoltre, emerge il dato dell'aumento della spesa corrente. La spesa primaria, come osservato nel Libro verde di Tommaso Padoa-Schioppa,

dimostrano tutto il loro limite: inefficace si è dimostrato il comma 507, peggio ancora la conseguente restrizione operata con il decreto-legge n. Finora, non emerge nessuna volontà di contenere la spesa pubblica, come ricordato dal collega Eufemi nel suo intervento. Invece, molto decisa è la volontà di aumentare le tasse per finanziare anche la spesa inutile e improduttiva. Non a caso, nulla del Libro verde è stato ripreso nella finanziaria. Per queste ragioni, il voto dell'UDC è contrario al disegno di legge di assestamento per il 2007. Colleghi del centro-sinistra, il Governo Prodi è percepito come un Governo contro gli italiani. La gente mi ferma per strada domandandomi quando lo mandiamo a casa. Siete soli contro gli italiani e, anche con questo voto contrario dell'UDC, rimarrete nel vostro isolamento. Non sappiamo quando ci sarà la resa, ma siamo sicuri che avverrà.

sottoposto all'approvazione di questo ramo del Parlamento, evidenzia un miglioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza di 4,2 miliardi di euro. Il saldo al netto della relazione contabile, e compreso anche l'impatto degli atti amministrativi,

ma non vi è dubbio che l'assestamento dimostri - e vorrei dirlo anche ad autorevoli esponenti della Banca d'Italia - che se è vero,

di aiuto, anche fiscale, ai ceti più deboli. Si è scelto di applicare nella sostanza quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della scorsa finanziaria. Tuttavia, emerge un dato importante:

chiedeva di destinare l'intero extragettito in riduzione del debito, posizione che, seppur con motivazioni diverse, è stata fatta propria dal Governatore della Banca d'Italia, anche se in questo modo non vi sarebbe stata alcuna opzione di crescita. Dall'altra

con tutti i limiti e con il carattere specifico dell'approvazione di un assestamento, complessivamente il Parlamento in questi mesi, prima discutendo la risoluzione sul poi la Nota di aggiornamento al 30 settembre, infine approvando questo assestamento, ha avuto la possibilità di dare un valore pubblico alla discussione sui conti pubblici, premessa per una discussione serena di una finanziaria rispetto alla quale la nostra sintesi politica è la seguente: sicuramente ci sono le condizioni perché, insieme ad una politica di risanamento, della quale dobbiamo tutti dare atto al Governo e al ministro Padoa-Schioppa,

*(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa meravigliosa estate romana, romana, illuminata oggi da una splendida giornata di sole, il Senato procederà ad approvare il bilancio dello Stato.

paradossalmente da parte della sinistra, quel magnifico film americano, pieno di profondi significati, dal titolo "Matrix". Il Senato, le istituzioni della Repubblica, le forze politiche stanno vivendo "Matrix", una realtà virtuale, piena di "bisteccone" pioggia a tutti e, soprattutto, alla povera gente, non volendo vedere la realtà vera, quella quella in cui gli umani sono sottoposti ad un continuo risucchio di sangue per produrre energia a vantaggio di pochi concentrati poteri. Cari colleghi della sinistra, quando uscirete da questo vostro "Matrix" nel quale è lo stesso vostro Governo a succhiarvi il sangue? Questa è la realtà che oggi il Senato vivrà, nella totale inconsapevolezza di che cosa sta votando in termini di bilancio dello Stato. Abbiamo avuto ieri la prova e la controprova che l'Aula non è in grado di conoscere i dati fondamentali della pubblica amministrazione e la loro rappresentazione numerica nel bilancio dello Stato.

pochi minuti fa, nella consueta inconsapevolezza dell'Aula, ha fatto una dichiarazione importantissima, che probabilmente verrà colta dal Fondo monetario internazionale, dall'Unione Europea, dall'OCSE e dalla Banca d'Italia sarà colta meno all'interno di questa Aula. Il collega Ripamonti ha affermato, finalmente, dopo più di un anno, la verità. ha detto, come chiunque potrà controllare nel Resoconto stenografico, che nel 2006 c'è stata una correzione di *deficit* di 1,3 punti di PIL,

che il *deficit* del 2006 è pari al 4,4 per cento, perché si utilizza il trucco contabile di aggiungere due poste di debito pregresso che non hanno niente a che vedere con il *deficit* di competenza.

perché è un'opinione che non condivido ma che rispetto in quanto almeno è trasparente, non subdola e mistificatoria come le posizioni di tante altre componenti all'interno della maggioranza e soprattutto del Governo. Egli ha affermato che sarebbe stato accanimento terapeutico accettare le linee guida dell'Unione Europea, che prevedono di ridurre di mezzo punto all'anno il *deficit*,

Contrariamente alle linee europee, il Governo, e Ripamonti lo ha chiarito, ha deciso di non rispettare le linee guida europee e di alzare il *deficit* pubblico cento quest'anno e al 2,2 per cento l'anno prossimo, rinviando al 2009 e al 2010 eventuali aggiustamenti per rispettare l'obiettivo di azzeramento del *deficit*. Questo è quanto avvenuto pochi minuti fa in Aula, un'operazione di chiarezza di cui do atto al collega Ripamonti.

allora da "Matrix", rendetevi conto che quei 25-30 miliardi che avete speso in più tra il decreto di luglio, il decreto del 1° ottobre e la finanziaria non servono affatto ad un'operazione di politica economica a vantaggio delle classi deboli e di chi più ha bisogno. Smettetela di pensare che l'opinione pubblica e i vostri elettori si accontentino delle bistecche fatte con i *software* e della realtà virtuale. La loro realtà autentica è quella della terza settimana del mese, alla quale molti non riescono ad arrivare ed è quella di considerarsi presi in giro e vilipesi con un aumento di 81 centesimi al giorno per le pensioni, di 41 centesimi al giorno per gli incapienti

questa gigantesca "Matrix" che si compie oggi ha un ulteriore elemento di paradosso. Mentre il Senato vota questo kafkiano assestamento di bilancio nel pieno dell'autunno e di una giornata piovosa (e mi fa piacere che almeno uno dei senatori della maggioranza si sia accorto che non siamo in estate e non c'è il sole), non c'è il sole), dentro le vostre manovre di politica economica è come dire che c'è il sole quando piove. Farò un'ultima riflessione, signor Presidente. Mentre oggi questa maggioranza, nella sua inconsapevolezza, evidentemente si diverte a vedere un film americano pieno di profondi significati per la nostra società attuale, con i controlli dei *mass media* e dei grandi poteri - questo è il messaggio di "Matrix" - dovremmo tutti uscire, insieme,

stravolti, un giorno sì e un giorno no, in un senso e nell'altro. Da Palazzo Chigi escono disegni di legge sul noto protocollo *welfare*.

l'eliminazione del tetto di 5.000 pensionandi per i lavori usuranti e la riapertura delle quattro finestre.

implicano un aumento del debito pensionistico del 25 per cento, che oscilla tra 200 e 250 miliardi di euro. Signor Presidente, mentre qui stiamo a discutere di 10 milioni, 20 milioni o altre cifre, contemporaneamente si sta decidendo un carico sulla generazione futura tra 200 e 250

si sta decidendo un carico sulla generazione futura tra 200 e 250 miliardi di euro in termini di debito pensionistico. Questo è ciò che sta avvenendo, signor Presidente, ed è per questo che annuncio il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

passato. È prassi, in questo caso, dichiararsi moderatamente contrari perché è un rendiconto della passata legislatura e fa, quindi, riferimento ad un bilancio e ad una finanziaria ben diversi:

perché, anche se è sempre difficile parlare di numeri in modo chiaro; tuttavia, con un po' di presunzione cercherò di farlo in quest'Aula. Il primo motivo

in finale un potenziale ricorso al mercato per 219 miliardi di euro e, quindi, un miglioramento delle previsioni rispetto al ricorso al mercato per 5 miliardi, anzi 5.330 milioni.

Cosa fa il Governo? Prende questi miliardi, li mette nella tabella e, a questo punto, migliora il saldo netto da finanziare. Ma dov'è la contraddizione che abbiamo cercato di riferire all'Aula e alla Presidenza nel momento in cui abbiamo presentato le nostre argomentazioni contrarie all'assestamento già nelle scorse settimane? Il problema è che questi 7 miliardi - che, sottratti i 3, diventano 4 - non migliorano il saldo netto da finanziare, perché i soldi dell'assestamento sono già stati spesi. Lei, signor Presidente, e l'Aula

nella buona sostanza. È stata introdotta la copertura per buona sostanza. Questo è il primo dei motivi. Qualora però non si volessero considerare questi motivi, che finiscono per essere motivi

poi venire a chiedere la fiducia. No. Noi siamo contrari, anche perché la fiducia è cosa seria e il vostro modo di governare - quello del Governo Prodi - non lo è.

di Luigi XIV, che sosteneva che l'arte di tassare è l'arte di spennare l'oca cercando di avere il massimo di piume con il minimo di starnazzi.

questo è più che evidente. Ma c'è di più e vogliamo spiegare l'arcano. Si dice che, gratta gratta, sotto la pelle di un russo si trova il cosacco. I postcomunisti oggi al Governo del Paese dicono di non mangiare più i bambini, però, gratta gratta, scopriamo che non vogliono mangiare i bambini, ma l'oca che hanno spennato, di cui non rimangono più né piume né penne, signor Presidente. Questo il Paese lo ha capito ed è questo il motivo per cui, interpretando il mandato

Ne ha facoltà. LUSI *(Ulivo)*. L'approvazione parlamentare del rendiconto generale dello Stato per l'ultimo esercizio finanziario concluso e dell'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso non costituisce un semplice adempimento contabile: esso rappresenta, invece, un passaggio cruciale per la valutazione non solo tecnica, ma anche e soprattutto politica, della credibilità e dell'efficacia dell'azione di Governo nella gestione finanziaria dello Stato. Questa è infatti l'occasione per una verifica concreta, da parte del Parlamento, della corrispondenza tra i risultati effettivi conseguiti nella gestione di riferimento e gli schemi di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa presentati dal Governo alle Camere. Ma la discussione sull'assestamento e sul rendiconto è anche la sede per acquisire gli elementi concreti necessari per individuare la cornice finanziaria entro la quale dovranno essere iscritte le politiche economiche della prossima manovra di bilancio. In tal senso, la duplice funzione, conoscitiva per un verso e giuridico-costituzionale per l'altro, di questi documenti di bilancio assegna loro un ruolo rilevante per il corretto funzionamento di una democrazia parlamentare che, quest'anno, si connota di una particolare importanza politica. Ad un anno e mezzo dall'inizio della legislatura, infatti, il quadro finanziario fornito dal rendiconto e dell'assestamento costituisce il primo e concreto riscontro dei risultati raggiunti dalle politiche del Governo Prodi sui fronti del risanamento dei conti pubblici e del riequilibrio allocativo. E sono proprio l'esito brillante di tale riscontro, da un lato (attestato da una *performance* dei conti pubblici di gran lunga migliore delle aspettative), e la ritrovata trasparenza nella rappresentazione del bilancio dello Stato, dall'altro, a restituire a questo passaggio parlamentare l'altra sua funzione propria, del tutto appannata nella scorsa legislatura: quella di consentire al Parlamento di conoscere il perimetro di riferimento della prossima manovra finanziaria e, dunque, di impostare il dibattito politico su presupposti finanziari certi e su basi conoscitive più solide rispetto al passato. A questo proposito, il cambiamento di passo delle politiche di bilancio in questa legislatura si annuncia come notevole anche sul piano sistematico e strutturale. Fin dal suo insediamento, l'attuale Governo ha infatti avviato un percorso pluriennale di riforma basato, per un verso, sulla ripresa del processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato e, per altro verso, sul completamento di un programma di revisione della spesa pubblica (la cosiddetta *spending review*), finalizzato a garantire la possibilità di riduzioni mirate e razionali delle spese e, quindi, una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse. L'obiettivo è quello di aggredire più efficacemente la rigidità della spesa primaria corrente, puntando a una struttura del bilancio che renda meglio valutabili gli effetti delle singole politiche di spesa attraverso un'aggregazione delle risorse pubbliche per missioni e programmi, sui quali concentrare l'esame e il voto parlamentare. Ma non meno rilevante, sul piano metodologico, deve ritenersi l'obiettivo di superare definitivamente la stagione dei tagli generalizzati e indiscriminati alla spesa delle pubbliche amministrazioni, recuperando lo spirito e il valore politico delle scelte gestionali che sottendono alle politiche di bilancio del Governo. La principale novità da registrare è, dunque, il materiale avvio di una nuova stagione nella gestione del bilancio, destinata in prospettiva ad incidere profondamente anche sulla qualità e l'efficacia delle politiche di intervento pubblico. Intanto, alcuni segnali positivi sul fronte della gestione del bilancio vengono già dal rendiconto per l'anno 2006. Per quanto riguarda le entrate finali, nel confronto con i dati gestionali del 2005, il miglioramento registrato nel 2006 rispetto alle previsioni è risultato di notevole entità. il positivo andamento delle entrate trovava un riscontro anche nel disegno di legge di assestamento per l'anno 2007. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica rilevato in quella sede - che sarebbe stato assunto di lì a poco a fondamento del quadro macroeconomico delineato nel DPEF 2008-2011 appariva già allora netto: il *deficit* tendenziale per il 2007 era indicato al 2,1 per cento del PIL, con un miglioramento di due decimi di punto, rispetto al livello previsto dalla "relazione unificata" del marzo 2007. È stato, dunque, il netto miglioramento della *performance* dei nostri conti pubblici, rilevato a metà dell'anno, a permettere nel luglio scorso la realizzazione di una significativa manovra redistributiva - realizzata con la conversione in legge del decreto-legge n. 81 - finalizzata a destinare nuove risorse, da un lato, al sostegno delle categorie sociali più deboli con l'adeguamento delle pensioni minime e, dall'altro, al finanziamento di interventi per lo sviluppo. A finanziare quel provvedimento - che avrebbe determinato un innalzamento delle stime di indebitamento del 2007 per circa 0,4 punti percentuali di PIL, peraltro coerente con il raggiungimento degli obiettivi concordati con la Comunità europea attraverso il Patto di stabilità e crescita - era stato proprio il cosiddetto tesoretto registrato dal disegno di legge di assestamento per il 2007. Si trattava di circa 7,4 miliardi di euro di maggiori entrate, ascrivibili in larga misura al comparto tributario: 3,3 miliardi di euro di maggiore gettito derivanti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, 1,6 miliardi di euro di maggiore IVA e circa 1,2 miliardi di euro di IRES. In quel contesto, il risultato complessivo dell'assestamento di bilancio 2007 evidenziava un miglioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza di ben 4,2 miliardi di euro. bilancio degli emendamenti correttivi dei saldi, con i quali si è almeno in parte recepito l'effetto sui conti pubblici delle autoliquidazioni, quel *trend* positivo di evoluzione dei conti pubblici rilevato nel giugno scorso non solo appare confermato, ma risulta perfino accentuato nella sua portata complessiva, al punto da assorbire pressoché integralmente gli effetti espansivi del decreto-legge Con una correzione al rialzo del *surplus* delle entrate, pari a circa 6 miliardi di euro, e una ulteriore riduzione delle spese per circa 2 miliardi di euro, il tesoretto risulta dunque a tutt'oggi ricostituito quasi integralmente, per un ammontare di circa 8 miliardi di euro. Sarà il Governo, attraverso la Nota di aggiornamento al DPEF, ad indicare l'entità degli effetti strutturali di questa correzione, destinati a proiettarsi sugli esercizi finanziari futuri. Tuttavia, signor Presidente, l'origine e la natura di questo eccezionale risultato di bilancio possono già chiaramente identificarsi in alcune delle scelte strategiche compiute dal Governo fin dall'inizio della legislatura. Esso deve ritenersi, infatti, in larga parte ascrivibile alle politiche di emersione della base imponibile e di miglioramento della *tax compliance* avviate dal Governo fin dall'inizio della legislatura. Anche la ripresa della crescita economica ha tratto beneficio dall'azione dell'Esecutivo, in particolare nel campo delle liberalizzazioni e degli interventi di potenziamento delle infrastrutture. Invertendo l'orientamento delle politiche tributarie attuate nei cinque anni precedenti, il Governo Prodi ha inserito la lotta all'evasione fiscale tra gli obiettivi strategici della sua azione, con ciò riconoscendo l'urgenza di incidere drasticamente su uno dei fenomeni che più pesantemente pregiudicano la qualità e la sostenibilità del nostro sistema economico. L'Italia si colloca, infatti, tuttora ai vertici delle classifiche per livello di evasione fiscale tra i Paesi dell'Unione Europea, con un'economia sommersa compresa tra il 16,6 per cento e il (cui corrisponde una perdita di gettito valutabile in circa 200 miliardi di euro l'anno). Nessuna seria politica di sostegno allo sviluppo può dunque prescindere dalla necessità di ristabilire durevolmente l'equità sociale e le corrette condizioni di concorrenza tra i soggetti economici attraverso politiche strutturali di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. I risultati conseguiti dal Governo in questa prima fase della legislatura dimostrano non solo che tale strada può essere imboccata con successo, ma che essa è il necessario presupposto all'adozione di politiche di contenimento della pressione tributaria in favore dei contribuenti più bisognosi e più leali. Non a caso, fin dalla legge finanziaria per il 2007, al comma 4 della stessa, il Governo si è impegnato a destinare in via prioritaria le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale laddove permanenti ed eccedenti gli obiettivi di risanamento - a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF 2007-2011, nonché alla progressiva riduzione del prelievo tributario a carico delle famiglie, in particolare di quelle numerose o incapienti, e dei soggetti economicamente più deboli, quali i giovani precari e gli anziani. 2008-2011 e la risoluzione parlamentare approvata al termine del suo esame hanno poi ulteriormente qualificato tale impegno, indicando come prioritari gli interventi di riduzione del carico fiscale sulla casa da realizzarsi attraverso l'abbattimento dell'ICI sull'abitazione principale, l'adozione di un sistema di tassazione separata per i redditi da locazione e il riconoscimento di detrazioni fiscali per i canoni di locazione. Il positivo andamento dei conti pubblici, certificato dall'assestamento per il 2007 e confermato dall'emendamento correttivo del Governo, inquadra oggi quegli impegni in una prospettiva finanziaria finalmente concreta, legittimando le aspettative del Paese per un nuovo corso di politica fiscale che meglio corrisponda alle esigenze di giustizia sociale e di sviluppo delle famiglie e delle imprese. D'altra parte, non è solo alla politica delle entrate che questo Governo ha affidato il risanamento. A dimostrarlo sono gli stessi documenti di bilancio oggi in discussione. Se il rendiconto 2006 evidenzia un miglioramento della spesa finale, con un risultato di gestione inferiore per circa 12 miliardi di euro rispetto alla previsione, l'assestamento indica in circa 2 miliardi di euro la correzione in diminuzione della spesa complessiva per il 2007, con ciò attestando un significativo recupero della capacità di controllo del bilancio anche sul lato delle uscite. In definitiva, il risultato complessivo che emerge dal rendiconto 2006 e dall'assestamento di bilancio 2007 evidenzia un netto miglioramento di tutti i saldi di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa: dal saldo netto da finanziare all'avanzo primario, che conferma una netta ripresa di quota dopo l'erosione subita durante la scorsa legislatura. Ma l'aspetto più rilevante dei documenti in esame è il quadro generale di finanza pubblica che da essi emerge, a partire dalla riduzione dell'indebitamento netto.

ai 2,1 punti percentuali di PIL registrati al momento dell'emanazione del decreto-legge n. 81, con un risultato che - in assenza della manovra espansiva del giugno scorso - potrebbe oggi attestarsi al di sotto del 2 per cento di PIL, a un livello largamente più basso di quanto imposto dai vincoli comunitari. Il margine che i documenti di bilancio oggi all'esame del Senato delineano per la prossima manovra finanziaria è, dunque, non solo in linea con gli impegni assunti in sede europea, ma anche pienamente compatibile con un percorso congiunto di sviluppo, equità sociale e risanamento finanziario. Esso attende la prossima legge finanziaria per essere proseguito e accelerato, in continuità - si auspica - con quella logica di rifiuto della strategia dei due tempi (il tempo del risanamento e il tempo dello sviluppo) affermata dal Governo fin dal primo DPEF presentato alle Camere in apertura di legislatura, quale obiettivo e assieme presupposto per una crescita elevata, duratura ed effettivamente sostenibile. È con questo spirito e secondo tale auspicio, signor Presidente, che annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo.

Presidente, come parlamentare vorrei esprimere disagio e forte riserva nei confronti della decisione assunta due giorni fa dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione in materia di eutanasia. Si criticano, spesso con ragione, quei politici che oltrepassano i confini della propria competenza ed esprimono valutazioni su decisioni giudiziarie che magari non conoscono. PRESIDENTE. Invito i colleghi che

ma questa pronuncia della Corte di cassazione, la n. 2174/08 del 16 ottobre 2007, pone di fronte ad una dinamica esattamente speculare. Nel momento in cui il Senato, e la Commissione Sanità in modo particolare, approfondisce da oltre un anno il tema del testamento biologico e delle dichiarazioni anticipate di volontà di trattamento, con un dibattito sofferto e serrato attraverso il giudice di legittimità interviene e fissa principi, non esclusivamente di diritto, fondati sulla legislazione vigente. Ho qui copia integrale di questa sentenza e vorrei capire su quale norma di legge in vigore si fondi, per esempio, una affermazione di questo tipo: «Il giudice deve negare l'autorizzazione,

quale sia la norma di diritto vigente che fonda un'affermazione di questo tipo: «Non vi è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino naso-gastrico costituiscono un trattamento sanitario».

affermare che i giudici sono chiamati per Costituzione ad applicare la legge e non ad inventarla. Signor Presidente, il tema che mi permetto di sottoporre alla sua valutazione non è quello di una disamina di una sentenza di Cassazione, evidentemente, ma quello del delicatissimo equilibrio di poteri che questa sentenza insieme ad altre pone all'attenzione, vale a dire il tema della creazione per via giurisprudenziale di istituti la cui elaborazione e il cui varo spetta al Parlamento

Il Senato non può essere indifferente rispetto a quest'invasione di campo e, soprattutto, non può ritenere le proprie scelte condizionate da principi affermati in modo così apodittico. Ritengo che sarebbe poco dignitoso che la nostra funzione fosse trasformata in quella di esecutori di improvvide e opinabili decisioni giudiziarie. Alla fine la decisione può anche essere quella di non varare da parte del Senato alcuna legge, ma il decoro del Parlamento esige che questa scelta sia responsabilmente assunta dalle Camere della Repubblica e non da una camera di consiglio.

il concetto di coma irreversibile è scientificamente superato, tanto è vero che il termine utilizzato abitualmente è quello di coma persistente o protratto, ma certamente non quello di coma irreversibile che

clinicamente superata e non utilizzata nemmeno nei grandi centri riveli quanto meno una precipitazione che non dà conto della complessità del problema.

è vivo e ha diritto di essere trattato e tutelato come una persona viva. Il bisogno concreto espresso da questo soggetto è quello della nutrizione parenterale. Questo è il tema forte - il famoso discorso del mettere

la senatrice Fiorenza Bassoli. Su questo punto stiamo discutendo. Non c'è chiarezza assoluta, accordo pieno, ma non vorremmo nemmeno essere scavalcati sul cuore del dibattito, cioè sul testamento biologico. L'altro punto cui fa riferimento il giudice è quello del consenso previamente espresso da Eluana attraverso la rete degli amici, il dialogo con la sua famiglia, rispetto al modo di volere essere trattata nel caso in

e la convinzione di voler, comunque, proteggere questa figlia, ma non abbiamo nessun elemento di certezza che garantisca quale fosse la volontà del soggetto, quando non era ancora paziente.

ieri sera, pubblicamente, il senatore Storace si è vantato che l'Assemblea non aveva dato alcun segno di solidarietà a Rita Levi-Montalcini. Avrei voluto ricordare le sue parole e chiederle il favore di ripeterle in in apertura di seduta. Rimpiango, pertanto, che questo non sia avvenuto, anche perché è stata detta una falsità molto grave, per le ragioni che riguardano il suo costituendo partito di fascisti. Purtroppo non ha potuto avere eco in Aula e mi dispiace, perché quel che è successo a me oggi non è mai accaduto. È per ragioni personali che si parla in coda ad una seduta,

essa detta condizioni astratte, non scientifiche e soggettive, e lo fa proprio per autorizzare l'interruzione alle cure di Eluana. Forse la Suprema Corte non si è resa conto della voragine che ha aperto, dichiarando che gli interventi terapeutici si potranno interrompere se il coma è irreversibile e se si dimostra che tale interruzione è quello che avrebbe voluto la paziente.

al secondo aspetto, pensare che un tribunale possa, attraverso testimonianze, desumere le eventuali intenzioni e in base a quelle decidere, è veramente aberrante. Vorrei che qualcuno qui alzasse la mano dichiarando pubblicamente che non ha mai cambiato idea, anche su questioni veramente molto rilevanti. Potremmo invece riempire l'Aula di testimonianze di persone che avevano deciso su questioni molto importanti, quali quelle della vita e della morte, e che poi, una volta che si sono ammalate o si sono trovate in condizioni del tutto diverse, hanno completamente completamente cambiato idea. Per Eluana, tra l'altro, non si tratta di staccare una spina, ma di eliminare un sostentamento di base: l'acqua e il cibo.

Tra l'altro, sapendo benissimo che queste persone soffrono, con molta compassione, diamo loro della morfina per non farle soffrire. Termino, signor Presidente, ricordando che i giudici non possono introdurre o avallare, attraverso proprie sentenze, atti di eutanasia. Non spetta a loro definire cosa sia l'accanimento terapeutico e quando esso ricorra: spetta alla classe medica. Né possono pensare di soffiare sul collo del Parlamento, per arrivare appunto alla questione del disegno di legge sul testamento biologico. Tutto questo atteggiamento da parte dei giudici non fa altro che avvelenare un clima

tutto il nostro disappunto, ma anche la nostra forte preoccupazione per questa invasione di campo. I poteri e le competenze vanno assolutamente distinti e questo la storia ce lo insegna. *(Applausi dai Gruppi*

del senatore Mantovano - fuori dalla legge. Secondo il Vaticano (mi riferisco agli articoli usciti su «L'Osservatore Romano» e alle dichiarazioni rese, in particolare, da monsignor Betori, ma anche dal cardinal Barragan), sarebbero sentenze emesse da un gruppo di amorali. Dissento radicalmente su queste due affermazioni. Trovo francamente inopinata, signor Presidente, anche l'ultima sollecitazione fatta al Senato della Repubblica dalla collega Bianconi, che la sollecitava addirittura a emettere a nome del Senato una specie di ingiunzione alla Corte Corte di cassazione. La sentenza dice una cosa semplice: il paziente ha, attraverso un suo pronunciamento, cioè un testamento biologico in qualche modo reso noto ad altre persone, il diritto di scelta sulla sua fine. Capisco che chi pensa che la vita appartenga a Dio, ad un Dio al quale crede, per essere più precisi, non possa in alcun modo condividere questa scelta, ma penso anche che questa scelta vada assolutamente riaffermata da parte di chi non ha un Dio al quale conferire la propria vita. In verità, la sentenza, che è meditata e argomentata secondo i princìpi di dottrina del nostro ordinamento, a cominciare da quello costituzionale, fa esplicito e implicito riferimento all'articolo 13, all'articolo all'articolo 32, ma anche, implicitamente, all'articolo 20 della Costituzione. Nel momento in cui la gerarchia vaticana invita cittadini italiani che esercitano funzioni pubbliche a rispettare, prima di ogni cosa, nell'esercizio della loro pubblica funzione, il loro precetto di fede, in quel momento essa invita cittadini italiani alla violazione dell'articolo 20 della Costituzione repubblicana. Penso che ci troviamo di fronte ad un problema enorme, che però è sempre lo stesso, ed è l'invadenza dell'azione nella sfera pubblica da parte della religione o di una fede religiosa. Questo è un fenomeno che avviene ad Oriente con l'Islam, ma anche ad Occidente, ossia nel nostro Paese, per iniziativa della Chiesa cattolica romana. Penso che questo non sia accettabile, perché siamo in presenza di una palese violazione di un principio di democrazia e di libertà che si chiama laicità. Siamo altresì in presenza di una palese violazione di quel rispetto per il pluralismo dei valori che è proprio delle società multiculturali del nostro tempo, che viene letteralmente spianato da questa pretesa dottrina

a proposito del relativismo della Chiesa cattolica di Roma, a partire almeno dal 1534. Noi siamo il Parlamento della Repubblica. Un potere dello Stato, cioè la Corte di cassazione, ha emesso una sentenza rispettando quel principio di laicità e contrastando implicitamente quel finto riformismo magari proprio di un partito nato da poco e non a caso silente in quest'Aula, che, a proposito dei diritti degli omosessuali o delle coppie di fatto, della concezione della famiglia, dell'interruzione di gravidanza e della fecondazione assistita stende un velo di silenzio e di oscurantismo, che dovrebbe coprire con il buio le ricerche scientifiche e le loro applicazioni pratiche, che potrebbero alleviare la condizione umana e di vita di milioni di persone.

che non ritiene la sua morale inferiore a quella dei credenti. Quella della Corte di cassazione è una sentenza di civiltà, che dovrebbe onorare la nostra democrazia, alla quale ci dovremo attenere e dalla quale dovremo trarre incoraggiamento e impulso per legiferare nel nome della vita e della tutela del diritto della laicità e della libertà delle persone.

Presidente, intendo porre l'attenzione non tanto sull'invadenza della Chiesa nei confronti dello Stato, qual è stato il senso e il significato dell'intervento di chi mi ha preceduto. Vorrei piuttosto fare riferimento a una sentenza, quella dei giudici, che entrano nello specifico di un diritto a vivere o diritto a morire. Entrerò nello specifico per esprimere quel senso di forte disapprovazione verso quanto disposto da questa recente sentenza della Cassazione Cassazione che scuote le coscienze, che solleva molteplici perplessità. Il compito della magistratura e dei giudici è quello di dare esecuzione alle leggi che ci sono, non di forzarle o di orientarne un'eventuale approvazione. rappresenta un fatto grave. Per la prima volta la Suprema Corte sancisce che la morte può essere considerata un diritto. Nella fattispecie, decide che è meglio per un essere umano morire, anziché continuare a vivere.

Dietro a questioni come il diritto a morire "dignitosamente" si nascondono cambiamenti della nostra vita che implicano la perdita di quello che era considerato il più sacrosanto dei diritti umani: il diritto alla vita, un diritto che andava affermato in qualsiasi condizione essa si presentasse. Allora, non è accettabile questo richiamo al pluralismo dei valori, che ad ogni piè sospinto sembra levarsi, contro l'ingerenza della Chiesa - questa invadenza pervicace - e che viene introdotto con la sentenza che tenta di trasformare l'essere umano da creatura a creatore e controllore sia nel momento che nelle modalità della nascita e della morte. Insomma, vogliamo in qualche maniera rifuggire dalla logica dei cosiddetti casi disperati, ai quali sembra voler indulgere non solo la stampa, ma anche altri organi dello Stato, per cercare di indirizzare verso scelte cosiddette buoniste, determinate da speciali emozioni, anche un eventuale intervento legislativo. Riteniamo che la sentenza sia stata inopportuna e abbia, in qualche maniera, costituito davvero un'inutile ingerenza nelle prerogative del Parlamento. È vero che l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto di rifiutare le cure, ma la Carta costituzionale afferma anche un altro diritto: la tutela e l'inviolabilità del bene della vita, quale valore fondamentale del nostro ordinamento. Il rifiuto dei trattamenti sanitari non può essere essere esteso anche all'idratazione e all'alimentazione: far morire di fame e di sete una persona, perché in coma, credo equivalga ad un accanimento - se volete - non terapeutico, ma umano. Mi rivolgo a lei, signor Presidente del Senato, affinché possa vigilare e garantire l'autonomia della Commissione e del Senato, perchè possa davvero essere immune da ogni tentativo di ingerenza o di pressione esterna, affinché venga salvaguardato quel sottile equilibrio di compiti, ruoli e poteri che riguardano il Governo, il Parlamento e la magistratura. Nella fattispecie, la Commissione e quest'Aula hanno il diritto di poter legiferare

anche perché è da un anno e mezzo che stiamo discutendo del tema del testamento biologico (so che lei, Presidente, ha le sue opinioni maturate sulla base di esperienze). C'è un dibattito importante in corso. Parallelamente ce n'è un altro sulle cure palliative, perché da una parte si pensa di uccidere i pazienti, ma c'è anche qualcuno che pensa che i pazienti vanno curati;

mai non sia stato considerato, per esempio, l'articolo 36 del codice di deontologia medica, che prevede il divieto di eutanasia attiva o passiva.

sull'istigazione o aiuto al suicidio, a proposito del quale anche lo strumento del consenso viene individuato come attenuazione della pena? Chi oggi può oggettivamente dire che una frase detta in un contesto passato può costituire una volontà inequivocabile in futuro? Chi di noi non ha detto ai propri figli: «Ti ammazzerei» oppure «Mi hai fatto tanto arrabbiare che fosse per me ti strozzerei»? Questo significa che un'intenzione

in cui si diceva che lo Stato poteva decidere quale vita era degna di essere vissuta e quale indegna di essere vissuta. Chi stabilisce questo principio?

non sta in piedi. Chi oggi può dire che questo tipo di vita vale meno di un'altra? Come facciamo a dire questo? Ciò significa che c'è una vita da cui magari possiamo espiantare gli organi

il Senato non debba essere *testimonial* né di una campagna contro la corruzione né di una campagna in favore della corruzione. Tra l'altro, mi piacerebbe che chi crea manifesti del genere (questo, era peraltro, firmato da una forza politica non rappresentata in Parlamento; non rileva qui dire se sia di destra o di sinistra, perché ritengo che questi comportamenti siano condannabili ed esecrabili indipendentemente da chi li pone in essere),

delle persone che ritiene corrotte o che sia stato accertato essere corrotte. Certo, è invece più semplice fare così, è più facile gettare fango sull'istituzione nel suo complesso, anziché prendersela con chi effettivamente ha le sue responsabilità. di un fatto gravissimo, che offende soprattutto le persone oneste, quelle che non sanno come difendersi. Signor Presidente, non parlo mai della mia onestà perché la ritengo un prerequisito della mia vita politica come della mia vita privata e ritengo che ciò valga per moltissime

Non entro nel merito della vicenda Storace, sulla quale ho una mia personale opinione, perché - ripeto - ritengo che la misura debba essere il modo con cui esercitiamo il nostro ruolo istituzionale. Ma il senatore Colombo ha affermato che il senatore Storace sta ricostituendo il partito fascista: lo ha testualmente affermato poco fa in quest'Aula,

La ringrazio, senatrice Allegrini, perché ha toccato un punto serio, sul quale bisogna riflettere ed operare. Appena ho avuto notizia di questo manifesto, il Senato ha provveduto ad interessare il questore di Roma,

operazione assolutamente inaccettabile e diffamatoria. Procederemo poi con i passi che riterremo necessari. **Sulla

più nutrita, ma credo che sia in ogni caso importante lasciare una testimonianza in quest'Aula. Voglio anzitutto apprezzare, signor Presidente, la posizione che ha assunto in merito al supposto richiamo della legge elettorale dal Senato alla Camera. Credo che se la legge elettorale al Senato ha un momento di stasi non è perché il Senato non lavori e i colleghi della Camera siano più bravi, più celeri, più attivi, ma perché vi sono questioni politiche che vanno risolte sul piano politico presso

che viene contrabbandata come una riforma che corregge il sistema istituzionale, venendo incontro alle necessità dei nostri tempi. Addirittura si è detto (ma qui si tratta solo di una enfatizzazione

ricordare (ma lo faremo in altra sede) a tanti colleghi che hanno sostenuto il presidenzialismo, il premierato forte e così via e che oggi magari, forse non avendo letto la riforma, ritengono che essa vada in quella direzione. Ma a me di questa riforma preoccupa la parte dedicata al Senato della Repubblica. Presidente, qualche collega - forse per ironia o in quanto preso da un *lapsus linguae* - ha parlato di riforma pensionistica. Sì, la riforma pensionistica dei senatori. Quella riforma prevede un Senato assolutamente non rappresentativo - lei l'avrà letto e sa il il Senato a che livello viene ridotto - e questo lo dico per stigmatizzare sia il punto di opportunità politica

gli esponenti dei partiti erano senatori, proprio perché il punto fondamentale della riforma era la questione del Senato federale, ed è evidente che il Senato federale deve essere per primo condiviso da chi dovrà subirne sul piano elettorale ed istituzionale le conseguenze sotto tanti profili. Allora, credo, signor Presidente, che sia anche sua responsabilità e suo ruolo stigmatizzare un simile atteggiamento, che porta poi necessariamente a

per rispetto della carica che ricopro, oggi ho detto che sono sempre pronto ad approfondire le questioni.

Lo scientismo in queste situazioni non ci aiuta nella risoluzione dei problemi, ma semmai a complicarli o a trovare soluzioni sbagliate. La soluzione in questo caso la si trova sicuramente dentro il progresso della scienza, ma la si trova dentro una risposta umana, perché è l'uomo al centro del progresso scientifico, è l'uomo al centro del mondo, non è la scienza stessa. Quindi, bisogna riportare ogni elemento alla propria dimensione. Noi siamo dentro una dimensione umana della nostra vita, la scienza ci aiuta a migliorare la dimensione umana, ma non è la dimensione umana ad essere dedicata al progresso scientifico. Peraltro, è difficile,

questione ci ha messo 60 pagine per spiegare un concetto, quindi la Cassazione qualche complessità l'ha sicuramente incontrata. Sifa anche fatica a definire cos'è un coma irreversibile: lo sappiamo che è difficile definire il coma irreversibile, quindi dire "staccate la spina quando il coma è irreversibile" è una definizione molto generica ma di difficile definizione anche scientifica oltre che umana. Sicuramente non possiamo accontentarci di dire che la Corte di cassazione ha invaso l'ambito legislativo, perché è anche un problema nostro e poiché noi siamo l'ambito legislativo siamo noi a dover entrare nel merito della questione. Dobbiamo farlo con più decisione di quanto abbiamo fatto finora. Probabilmente, anzi sicuramente, c'è un'esigenza in questo Paese di interpretazione

Questo oramai è un percorso che abbiamo iniziato e che, inevitabilmente, dobbiamo concludere, altrimenti verremmo meno al nostro compito di legislatori, qualsiasi sia il nostro credo, la nostra fede politica, l'idea che seguiamo: abbiamo il compito

ai pazienti, ai parenti dei pazienti e anche agli operatori medici che si trovano ad affrontare condizioni complesse spesso senza armi o esponendosi essi stessi al pericolo.

di quando e come sia giusto morire, ma anche di come sia giusto vivere davvero dignitosamente fino all'ultimo momento della propria vita.

ha iniziato a discutere di testamento biologico - anzi, meglio, di dichiarazione anticipata di volontà - ben prima dei casi eclatanti che hanno evidenziato all'opinione pubblica la questione.

dei soggetti. Quindi, no all'accanimento terapeutico, ma no anche all'abbandono terapeutico. Su questi due princìpi mi sembra che la Commissione stia lavorando saggiamente e saldamente. Non c'entra l'eutanasia,

che la Corte non invada il campo legislativo; non c'è da porre limiti e paletti ad una Corte di cassazione che svolge il suo mestiere, cioè quello di giudice di legittimità

la competenza istituzionale è di quell'organo che l'ha espressa: noi ne dobbiamo tenere conto e non il contrario, se vogliamo davvero rispettare la divisione dei poteri e l'ambito in cui ciascuno è chiamato ad operare.

non può operare saltando questi due princìpi, dall'altro ricordandoci l'urgenza del provvedimento. È chiaro, infatti, che accertare la volontà sarà più semplice se avremo un atto di dichiarazione di volontà anticipata, ma la Corte afferma che anche in assenza di questo atto formale si possono accertare gli elementi

Signor Presidente, anch'io voglio esprimere la valutazione mia e del mio Gruppo sul dibattito che si è aperto dopo l'intervento del collega Mantovano.

La sentenza della Corte, come ha efficacemente ricordato la collega Boccia poco fa, non interviene nel merito della vicenda ma richiama i giudici di merito a tenere conto delle volontà e degli orientamenti espressi dalla persona prima che entrasse nello stato di coma irreversibile e nella fase vegetativa, per poter prendere una decisione di merito. Ciò testimonia l'urgenza di una legge sul sul testamento biologico che sia ispirata ai princìpi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione, nel quale si afferma esplicitamente, in maniera

Sono questi i cardini ai quali bisogna ispirarsi. L'eutanasia non c'entra assolutamente nulla con questa vicenda: il punto è esattamente come il Senato, che da un anno e mezzo è bloccato nella discussione dei vari provvedimenti di legge, riesca a riesca a fare fronte ai bisogni, alle esigenze, che come si vede drammaticamente già in questo anno e mezzo sono emersi e sono stati portati all'attenzione dell'opinione pubblica. È un nostro

alla luce di quanto avvenuto e anche di questa sentenza della Corte di cassazione, dovrebbe spingere in maniera seria e serena a entrare nel merito e

Signor Presidente, a proposito della sentenza della Corte di cassazione, sulla quale è stato introdotto dal collega Mantovano il dibattito nella nostra Aula, debbo dire che io non vedo alcuna invasione di campo da parte della Corte stessa. Sono decisamente contrario rispetto all'invito, formulato dalla collega Bianconi, affinché il Presidente del Senato compia un passo per esprimere preoccupazione e ostilità rispetto alla pronuncia della Corte Siamo di fronte a una sentenza che sviluppa un ragionamento giuridico complesso e articolato,

valuta il principio, su cui tutti siamo - a parole - d'accordo, dell'autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari e della necessità del consenso informato. Da questo

e la sospensione dei trattamenti sanitari non è stata giudicata atto penalmente rilevante. Se la Corte di cassazione dice

piano giuridico, costituzionale e anche parlamentare. Ma abbiamo noi il diritto di impedire ad un magistrato, nel valutare un precedente giudicato, di indicare per i giudici successivi - i cosiddetti giudici del rinvio - quali sono gli ambiti nei quali la valutazione futura dovrà muoversi, avendo il magistrato espresso un giudizio su una questione che viene sottoposta alla sua valutazione?

che esistono tra chi produce le leggi, chi le applica e la libertà di interpretazione della funzione giurisdizionale al massimo dei livelli, stabilendo

perché la dignità del Senato non si manifesta solo quando i manifesti sono ingiuriosi, ma anche quando si chiede al Senato di fare qualcosa che non può e non deve fare. Il professor Pompeo Biondi diceva in toscano «e non si pole e non si deve», vale a dire non si può e non si deve

come morire, se la vita non è più degna di essere vissuta in certe condizioni. Questo non è relativismo etico, ma significa vivere la realtà dei propri tempi e non ancorarla a parametri di un passato

garantire al senatore Angius, preoccupato di una verticale caduta di laicità nell'azione di un partito appena nato, che questa caduta di attenzione e di laicità non ci sarà. sarà. Sulla questione dei precedenti e sul diritto a non curarsi, come viene motivato dalle 60 pagine della sentenza, ci sono almeno 16 anni di lavoro dei giudici della Cassazione, della Corte costituzionale e così via.

nell'ultima sentenza, la centralità della figura del tutore nella tutela anche dei beni non materiali della persona interdetta, in questi casi della sua libertà e dignità personale. I 16 anni di lavoro dei giudici

all'appello del senatore Biondi - un intervento censorio del Senato nei confronti della magistratura, che non si è mai esplicitato nei 16 anni che ci sono alle spalle e che hanno fissato dei paletti, entro cui la legislazione

come un aiuto al difficile e lungo lavoro legislativo, che pur sta avvenendo nella Commissione sanità del Senato, che però mi auguro possa arrivare a quella sintesi laica di contenimento e di Governo dei molti valori in gioco,

cerca di criticare l'invadenza, come ha detto qualche collega, della Chiesa, si possa contemporaneamente confrontare

Colgo l'occasione in conclusione anche per fare un appello alla maggioranza. Sapete che l'opposizione ha dovuto ridurre enormemente gli emendamenti, in primo luogo perché quasi mai vengono accolti, in secondo luogo, strategicamente, per evitare che ci sia l'alibi dell'apposizione

che vogliono morire, come è stato detto qui, ma anche ai tanti che vogliono vivere i loro momenti fino alla fine e che oggi sono stati a lungo presi in giro, perché gli è stata promessa una struttura che praticamente non è presente in quasi tutto il territorio. Quindi cogliamo l'occasione, coerentemente con quanto affermato da tutti i presenti, per lavorare nella finanziaria al fine di realizzare ciò che di fatto doveva essere già realizzato da anni. Presidente, confidiamo nel suo aiuto.

La non negoziabilità di alcuni istituti è patrimonio di tutto il popolo italiano, a prescindere dalle interpretazioni che noi partiti ne facciamo. Se è vero questo, nel passato si era trovato un giusto equilibrio tra posizioni diverse, un equilibrio che è durato dalla Costituzione (dall'articolo 7 agli articoli 29-30 e successivi sulla famiglia) in poi. Perché vogliamo rompere questo equilibrio?

tutti in quest'Aula condividano (e mi sono un po' sorpreso di alcune affermazioni). Credo che, a partire da me, tutti ritengano che una vita in stato vegetativo permanente sia assolutamente una vita

credo si possa articolare in due aspetti. Il primo è stato sottolineato da tanti prima di me, e lo dico con semplicità. Non sono certo in grado di dare consigli di giurisprudenza al Presidente del Senato e non mi permetterei neanche; credo non ne abbia bisogno. Ritengo che il potere giudiziario in Italia sia legittimamente rappresentato da ogni singolo magistrato e quindi che non vi sia possibilità o spazio per fare dei commenti su ciò che è la sentenza di una Corte. Penso però che questa sentenza, come altre in questi anni, in questo e in altri Paesi,

senza nessuna implicazione nel merito delle sentenze, il percorso su questi temi è iniziato nelle aule dei tribunali. Non credo che quella sia la sede adatta. infatti che i magistrati siano felici di dover incidere su questi temi. Soprattutto, è chiaro che se si affida a un magistrato una decisione su di essi, spesso si avranno decisioni diverse. È evidente,

persone in stato vegetativo permanente non ricevono solo l'idratazione o la nutrizione, ma anche tante altre terapie. Nel caso di Eluana Englaro Englaro (prima di parlare sono andato personalmente a trovarla), ella riceve la terapia antiepilettica tre volte al giorno, altrimenti morirebbe per crisi epilettiche; riceve l'eparina, altrimenti nel giro di due o tre settimane morirebbe di tromboembolia polmonare; riceve altri trattamenti affinché il suo intestino possa continuare a funzionare. Il suo intestino, infatti, viene svuotato diverse volte al mese meccanicamente: ciò significa che la mano di qualcuno deve entrare nel suo retto retto e svuotarlo quando lei non riesce da sola. Tutto ciò ritengo sia assolutamente legittimo, come credo che ognuno di noi possa scegliere in piena libertà se vuole tutto quel supporto tecnologico, quel supporto umano e quelle risorse e possa dare indicazioni, così come altri

chi crede profondamente - e sicuramente mi iscrivo tra quelli - nell'autodeterminazione delle scelte e quelli che invece in proposito hanno dei dubbi. Penso che su questo tema dobbiamo arrivare a un confronto e a una sintesi prima in Commissione sanità e poi nell'Aula del Senato. Dobbiamo, insomma, decidere se vogliamo dare a tutti quei cittadini che lo richiedono, e ai medici che hanno detto più volte di sentire il bisogno di una legge in materia,

Signor Presidente, vorrei esporle il caso drammatico di Er Avni, un giovane dirigente del partito comunista turco, rinchiuso, nel silenzio generale, da anni nelle carceri di Bad'e Carros, in Sardegna. Il fatto è questo: il 1° aprile 2004 furono arrestati a Perugia due cittadini turchi e tre cittadini italiani, accusati dal Governo turco di aver costituito una cellula terroristica quale articolazione in Europa del DHKP, un'organizzazione solidale con i comunisti e le forze di sinistra turche e immessa da poco, in un modo improvviso e tutto da capire, nella lista nera dell'Unione Europea delle organizzazioni cosiddette terroristiche. L'operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla procura della Repubblica di Perugia, assunse una dimensione transnazionale coinvolgendo con rogatoria internazionale l'autorità giudiziaria olandese, belga, tedesca e greca, oltre che la stessa magistratura turca, la quale autonomamente dispose l'arresto di oltre 80 attivisti impegnati nel campo dei diritti umani e dell'informazione. Il 20 dicembre 2006 la corte d'assise di Perugia ha ritenuto responsabili di partecipazione all'organizzazione DHKP

che tutte le persone fermate in Turchia, appena sono comparse innanzi alla corte di quel Paese, hanno dichiarato di aver subito maltrattamenti e torture da parte dell'antiterrorismo e che in tal modo erano state estorte dichiarazioni ad alcuni arrestati; che, nonostante la richiesta di rogatoria e l'esecuzione di perquisizioni e sequestri all'estero, nessun provvedimento veniva assunto dalle autorità giudiziarie del Belgio, dell'Olanda e della Germania, seppur, secondo l'ipotesi degli inquirenti italiani, in tali Paesi avrebbe soggiornato l'intero gruppo dirigente del DHKP. che neppure le autorità olandesi assumevano alcun provvedimento nei confronti dei soggetti rinvenuti nelle sedi perquisite, nonostante, secondo gli inquirenti italiani, fossero gli autori delle comunicazioni ricevute da Er Avni a Perugia, e pertanto da identificare come il vertice dell'organizzazione. Consideriamo, signor Presidente, che la Turchia è il Paese che negli ultimi quaranta anni ha conosciuto il dramma e la violenza causata da ben tre colpi di Stato perpetrati dall'esercito, che l'ultimo golpe è avvenuto nel 1980 e la legislazione e la Costituzione di quel Paese sono ancora il frutto di quanto legiferato e stabilito dai militari al potere

ha evidenziato la permanenza di trattamenti inumani e degradanti cui sono sottoposti gli arrestati e i fermati, soprattutto se accusati di terrorismo, e che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato la Turchia per la pratica della *falaka*,

con cui dichiara che lo Stato turco mantiene l'impunità per i funzionari pubblici responsabili di torture ed uccisioni extragiudiziali. È proprio di questi giorni, inoltre, la notizia secondo la quale il Governo turco evoca l'intervento armato in Iraq, scoraggiato fortemente anche dagli USA. USA. In data 7 maggio 2007, il ministro della giustizia Clemente Mastella, su domanda del suo omologo turco, ha richiesto alla corte d'appello di Sassari, competente per territorio, la custodia cautelare in carcere di Er Avni, nonostante lo stesso fosse già detenuto in forza del titolo privativo della libertà emesso dalla corte di assise di Perugia. La scelta del Ministro della giustizia, peraltro, è stata motivata dal pericolo di fuga e, pertanto, dal timore che Er Avni, detenuto presso le carceri di Nuoro, potesse comunque sottrarsi all'estradizione. In considerazione di tutto ciò, signor Presidente, chiedo se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno attenersi a quanto accertato in sede di istituzioni comunitarie sulle violazioni commesse in Turchia in materia di diritti umani e conseguentemente, secondo quanto previsto dall'articolo 698 del codice di procedura penale, nonché dal diritto comunitario e internazionale, non concedere l'estradizione